La seduta è ripresa.

nonché per evitare, possibilmente, un eventuale ricorso alla Corte costituzionale, mettendo bene in evidenza che il riferimento all'articolo 2 della Costituzione

all'impossibilità di sacrificare unilateralmente, tra diritto alla vita e diritto all'autodeterminazione, uno dei due, e a garantire, da un lato, la libertà di coscienza del medico e, dall'altro, il vincolo per le strutture sanitarie. Quindi, l'emendamento rimette dentro la costituzionalità questo articolo 1.

hanno significato anche le norme di principio, come peraltro dimostrano le molte affermazioni di principio presenti, a partire proprio dall'articolo 1 del testo che stiamo esaminando e a partire dal concetto della indisponibilità della vita. Inoltre, signor Presidente, lei non può sospettare quale consenso avrebbe nel Paese l'approvazione da parte del Senato da lei presieduto, di una norma che afferma al primo comma

*(PD)*. Signor Presidente, anche qua, riteniamo che, se non altro, si possa lavorare di cesello; quindi, proponiamo di togliere la lettera *b)*, che recita: «riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza» come se, invece, il contrario accadesse o vi fosse qualcuno che in effetti volesse che accada. Chiedo per questo la votazione

Dire che la dignità del paziente prevale sulle esigenze scientifiche è dire una cosa che ha un senso; dire che la dignità prevale sull'applicazione della tecnologia e della scienza, o non vuole dire nulla, vuol dire che ci sono applicazioni della tecnologia e della scienza che, pur giovevoli per la salute, non possono essere messe in opera perché ledono la dignità della persona. E vorrei ricordare, a questo punto, che da parte della magistratura, in maniera molto pretestuosa, si disse che

Perché dico questo? Di recente Ernesto Galli Della Loggia, in un suo pezzo sul «Corriere della Sera», ha messo in evidenza come la Costituzione italiana non è disinteressata, neutra,

cioè dimostra concretamente di sentirsi protagonista e di intervenire per tutelare, riconoscere, garantire e proteggere i diritti fondamentali del cittadino. Come abbiamo visto, all'articolo 2, la Repubblica si impegna a difendere i diritti inviolabili, tra i quali viene annoverato il diritto alla vita. All'articolo 32, invece, la Repubblica, cioè il soggetto attivo, tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. Quindi, sottolineo con forza che nell'articolo 2 il diritto alla vita è definito inviolabile mentre nell'articolo 32 il diritto alla salute, cioè il diritto a vivere bene, come è tecnicamente definito in tutti i documenti, viene invece ritenuto fondamentale e quindi derogabile. Dove si annida la radice del diritto del paziente a rifiutare le cure? Secondo l'interpretazione dei nostri colleghi di centrosinistra, questa radice si rinviene nel secondo comma dell'articolo 32: i lavoratori preparatori ed il dibattito approfondito hanno sempre dimostrato che il secondo comma dell'articolo 32 si riferisce ad una tutela generalizzata degli interessi dei cittadini. Il "nessuno" di cui si parla è un'espressione che molto spesso si rinviene in Costituzione per dire che la norma è pensabile *erga omnes*. Se non fosse così, paradossalmente, cioè se la lettura del secondo comma fosse quella che propone il centrosinistra, nel senso che solo per legge può essere imposta una determinata cura, allora il famoso decreto Berlusconi sul caso Englaro doveva essere obbligatoriamente costituzionale, perché era la legge che interveniva su un singolo caso ad obbligare ad un determinato intervento. Ma ovviamente non penso e non credo che i nostri colleghi di centrosinistra vogliano ritenere che allora i Costituenti abbiano detto che ciascuno può rinunciare al proprio diritto, a meno che non si faccia una legge per il paziente di Capizzi,

Sennonché, a mio avviso, manipolando il significato della Costituzione e aggirandola, è invalso l'uso di dire che il medico ha bisogno del consenso del paziente. Non sono d'accordo con questa interpretazione, perché a mio avviso è soltanto un modo per scaricare di responsabilità il medico e di fatto mettere il paziente nella condizione di non potere, nel caso in cui dalla cura dovesse derivare un esito discutibile, far valere i propri diritti; tanto firma un consenso preventivo tra parti, che nonostante noi si pensi debbano essere informate, come sappiamo versano in una situazione asimmetrica. allora propongo di dire che il paziente può esprimere il dissenso e che il medico ha l'obbligo di informare? Perché intanto il medico deve informare su quello che propone; il paziente, nel momento in cui dissente, esprime sì il proprio dissenso informato, che ha un grande valore, ma obbligando il medico soltanto ad informare nella condizione di poter intervenire quando l'esito della cura dovesse essere per caso deleterio, gravoso o dannoso. Perciò ritengo che correttamente, in base all'interpretazione dell'articolo 32 non si possa parlare di consenso informato nel senso in cui lo ritiene anche la proposta di legge, perché questo, di fatto, danneggia il paziente. Il paziente deve essere informato come vedremo dai successivi emendamenti l'informazione deve risultare per iscritto. Dopodiché, se dissente, a quel punto deve esprimere il proprio dissenso per iscritto. È un'impostazione che apparentemente può sembrare più restrittiva ma, di fatto, tutela il paziente rispetto a tutti quegli interventi che non potrebbe più porre in essere nel momento in cui esprime il proprio consenso (e sappiamo che negli ospedali è invalso l'uso di dire: «Dai, metti una firma» e poi, alla fine, sappiamo che finisce come finisce).

speravo che questo invito al ritiro non mi fosse rivolto, però, rispetto a una richiesta così poderosa, comprendendo che la maggioranza cerca un'intesa con l'opposizione, solo in questo spirito, ritiro l'emendamento.

all'articolo 32 della Costituzione, perché così formulata tale lettera non risulta chiara. Partiamo dal presupposto che il principio

Non solo, nella parte che segue, si fa riferimento all'alleanza terapeutica tra il medico ed il paziente, ritenuta nel testo del relatore prioritaria e in grado di acquistare valore proprio in una fase di fine vita. Crediamo che l'alleanza terapeutica abbia sempre lo stesso valore. Anzi, deve valere allo stesso modo in qualsiasi fase della vita e non si può scrivere in una legge che in una determinata fase un principio etico assoluto come l'alleanza terapeutica

«impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 2, comma 4, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

«e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà

Presidente, in questa fase del voto volevo richiamare l'attenzione dell'Aula all'aggiunta che noi proponiamo dopo la lettera *d)* del comma 1

non c'è alcuna intenzione di mescolare - per così dire - le questioni relative all'eutanasia sotto qualsiasi forma con le questioni relative al testamento biologico. Sono tematiche completamente diverse e in questo senso viene proposta, appunto per evitare la confusione, la soppressione semplice in questo momento della lettera

del codice penale che vietano l'eutanasia; pertanto, visto che la confusione è stata fatta, a questo punto utilizziamola in altro modo per disciplinare e regolamentare per legge l'eutanasia, che

formulazione: «*e)* prevede che ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, è regolamentata in conformità agli articoli 13 e 32 della Costituzione». Più volte ci siamo posti il problema relativo all'eutanasia nel dibattito anche in Commissione e la risposta è sempre stata la stessa, cioè *niet*. Non basta dire no per cancellare un fenomeno; questo esiste, è sommerso

Stiamo facendo una battaglia forte per introdurre una buona legge sul testamento biologico; l'eutanasia è un'altra vicenda, non c'entra niente e il nostro voto è convintamente no rispetto all'emendamento

con l'emendamento 1.198 eliminiamo la parte ridondante e pleonastica che ricorda l'esistenza del codice penale e, a titolo personale, faccio la dichiarazione di voto a favore di questo emendamento che almeno riconosce il diritto alla morte dignitosa.

brevissima dichiarazione di voto a titolo personale. Se davvero dobbiamo ricordare l'esistenza del codice penale, vi chiedo di ricordare anche l'esistenza dell'articolo 583 583 e, quindi, delle lesioni personali gravi. Quando un medico mette le mani addosso a un paziente senza il suo consenso sta facendo una lesione personale grave. Chiedo

e poi dice che è vietata forma di eutanasia, di assistenza o di aiuto al suicidio), non essendo univoci questi riferimenti nel nostro ordinamento, provoca una mostruosa espansione del potere dei giudici e, quindi, determina un'incostituzionalità ai sensi dell'articolo 25 e uno strapotere degli organi giudiziari. Questo comma è stato ritenuto incostituzionale anche dal vostro Capogruppo in Commissione affari costituzionali della Camera, onorevole Calderisi.

Signor Presidente, desidero ringraziare il relatore e il Governo: è stato un parto difficilissimo, ma ce l'abbiamo fatta e quindi sono particolarmente soddisfatta.

1ª Commissione permanente, esaminato il testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando che non appare chiaro, all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 5, comma 1, il senso dell'espressione: "azienda sanitaria locale di competenza regionale". Si segnala inoltre, sempre all'articolo 5, comma 1, la possibile lesione delle competenze regionali in materia di assistenza e di organizzazione sanitaria. Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sull'emendamento 5.100, a condizione che l'espressione "d'intesa con la" sia sostituita dall'altra: "previa intesa in sede di", e che l'espressione "cui le Regioni si conformano nell'assicurare" con l'altra: "nell'ambito delle quali le Regioni provvedono affinché sia assicurata"; esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno dì legge in titolo, in riferimento all'articolo e 5.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 9.1, 9.6, 9.25 e 9.100

al comma 4), sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.269

*(PD)*. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione del relatore e del Governo, in particolare del ministro Sacconi,

una misura di trasparenza nei confronti dei cittadini e di semplicità per l'accesso a quello che i cittadini possono fare rispetto a una legge approvata. Quindi, qualunque sarà la natura della legge, si chiede semplicemente che possa essere resa disponibile sul sito Internet del Ministero della salute.

questione è, manifestamente, una norma manifesto nel senso che, con atti e comportamenti dell'Amministrazione, questa diffusione viene assolutamente garantita. Non si vede pertanto la ragione di dare forza di legge a comportamenti dell'Amministrazione.

sono improcedibili. Poiché non sono stati approvati emendamenti all'articolo 1 tali da modificarne il contenuto in modo sostanziale rispetto al testo proposto dalla Commissione,

mio intervento vale anche come dichiarazione di voto del mio Gruppo sull'articolo 1. Io tengo innanzitutto a ringraziare il senatore Nania per il contributo che ha portato al dibattito e per i chiarimenti che ha dato in merito all'equilibrio costituzionale che esiste fra l'articolo 2 e l'articolo 32. Ed è per questo che, quando noi facciamo riferimento all'uno, facciamo sempre riferimento all'altro. Posso dire, a titolo personale, di essere d'accordo con l'interpretazione che il senatore Nania dà dell'articolo 2 e di essere anche d'accordo sulla sua definizione di dissenso, che trovo più corretta. Tuttavia, questo articolo 1 è l'articolo che fissa il lessico della legge. E questo lessico è stato la ricerca di un equilibrio paziente, in alcuni casi anche di un compromesso, che ha portato noi a dialogare con le opposizioni e a trovare delle soluzioni che sono state ampiamente condivise. Poiché riteniamo che questa legge sia una legge di compromesso in senso nobile, come è inevitabile che sia quando si entra in questioni che sono quelle che concernono il testo che stiamo esaminando, riteniamo di non dover spostare l'equilibrio che abbiamo ricercato e di farlo nella consapevolezza che fissare il lessico comune è quello che ci potrà portare con più serenità a dividerci sulle soluzioni concrete nei prossimi articoli. Dunque, io prego il collega Nania di considerare il senso politico di queste osservazioni e di accettare il ringraziamento sincero che viene dal Gruppo. Chiedo inoltre ai colleghi dell'opposizione di apprezzare apprezzare questo sforzo di lealtà e questo senso che abbiamo voluto dare a questo articolo.

siccome prendo atto che ogni volta che si fanno le leggi si costruiscono anche i presupposti per vedere poi il contenzioso a me sembra un punto fondamentale che l'inviolabilità della vita sia un'inviolabilità che riguardi il proprio titolare. Mi sono meravigliato, perché prima mi era stato detto che su questo punto si poteva trovare un accordo anche perché ritengo che, non precisando che il diritto è un diritto inviolabile anche da parte del suo titolare, noi di fatto, rispetto ad uno sforzo che è stato fatto in questa legge di definizione complessiva della materia, teniamo in piedi e diamo la possibilità, successivamente, di mantenere un equivoco che ci può portare in futuro a vedere nuovamente ripetersi tanti casi Englaro. Se noi scriviamo che si attua l'articolo 2 della Costituzione, che giudica inviolabile la vita, e lo scriviamo nella legge in modo chiaro, stabilendo l'inviolabilità della vita anche da parte del suo titolare, noi avremo fatto un passo in avanti molto significativo e molto importante. Pertanto io, proprio

è quello fondamentale di questa legge. Avremmo voluto che ci fossero la possibilità e il modo di riprendere anche qui in Aula un confronto che pure c'è stato

la legge manchi, perché non si spiega con la necessaria chiarezza il perché della necessità di legiferare su questo tema. la necessità nasce dal progresso medico e scientifico, che ha cambiato la nostra percezione di vita e di morte, ma che ha anche cambiato il significato e il senso della parola "salute": è cambiato, di conseguenza, il rapporto con il medico e con la realtà circostante. Pertanto, è necessario che la legge, proprio per queste ragioni,

A me pare che questa possibilità venga a mancare, in quanto in quest'articolo si affermano e contemporaneamente si negano i principi costituzionali, principi costituzionali, che riconoscono appunto il diritto di esprimere il proprio consenso alle cure a cui si è sottoposti.

Forse perché questo tema del consenso informato sarebbe stato contraddetto dalla priorità che date nello stesso comma Allora, costruire un'alleanza terapeutica significa costruire un percorso condiviso, non un atto basato su una posizione di predominio da parte del medico, come appare nella priorità che date in quest'articolo. comunque che quest'alleanza che si deve creare tra medico e paziente non sia peculiare solo nel fine vita: è stato detto in diversi interventi svolti in Aula

Riteniamo anche sbagliato richiamare nella legge il codice penale, che vieta l'eutanasia, nonché l'assistenza e l'aiuto al suicidio. Quando la legge ha iniziato il suo *iter* è stata fatta una scelta chiara: non si doveva discutere nessun testo che facesse riferimento all'eutanasia. Su questo noi siamo stati fermi in tutto il dibattito in Commissione ed anche in Aula, come è stato detto dal senatore Bianco. Credo quindi che, per tutte queste ragioni, sia importante ribadire, anche per l'aggravamento nella definizione di consenso informato e di accanimento terapeutico, in seguito all'approvazione di alcuni emendamenti*...* Colleghi, così non possiamo continuare. Purtroppo, se dovessi sospendere la seduta per mezz'ora per poi riprendere, non chiuderemmo i nostri lavori nella serata di giovedì. Vorrei quindi significarvi questo aspetto: se questa Presidenza, durante queste giornate, per ricondurre l'Assemblea a compostezza, dovesse essere costretta più volte a sospenderne i lavori, il calendario dei lavori, approvato all'unanimità dai Capigruppo, non potrebbe obiettivamente essere rispettato. Se è interesse dell'Assemblea mantenere fede

Ve ne è anche uno di minore rilievo, ma quello più importante riguarda l'invenzione - letteralmente - del concetto di indisponibilità. Già sul concetto di inviolabilità si potrebbe ragionare, perché qui il collega Nania ha valentemente "stiracchiato" l'articolo 2 per dimostrare che la vita è un diritto inviolabile e indisponibile; ma in realtà l'articolo 2 parla dei diritti inviolabili, non del diritto alla vita. Ricordo che il termine "vita" compare in Costituzione per la prima volta all'articolo 38, laddove si parla dei diritti del lavoratore a veder salvaguardata la vita dagli infortuni sul lavoro. Il diritto alla vita è un diritto non scritto; sarà sicuramente compreso all'interno dei diritti inviolabili, ma non se ne può trarre una conseguenza geometrica obbligata e trasformarla in un postulato da cui non si può tornare indietro. Ma non è tanto sulla questione dell'inviolabilità che mi voglio soffermare, Questo concetto della indisponibilità è letteralmente inventato e sarei curioso di sapere chi ne è l'autore, perché viene fuori da non si sa dove.

Cos'è questa storia della indisponibilità? Perché si deve ragionare in questi termini? In realtà, c'è un sottofondo, piuttosto subdolo, abbastanza ipocrita da non volersi dichiarare per cui si sostiene che la vita è indisponibile per chi la vive e il sottofondo nascosto è che, se la vita è indisponibile per chi la vive, è disponibile per qualche autorità superiore. Queste autorità superiori possono essere solo due: o Dio o lo Stato. Nella legge non si può scrivere che la vita è indisponibile perché è disponibile per Dio; saremmo all'apertura dello Stato teocratico e nessuno osa tanto. Si deve allora dichiarare che è indisponibile perché - sotto sotto, non dichiarandolo - è disponibile per lo Stato. Solo lo Stato può determinare qualcosa in tale campo. Questo è un punto insidioso, perché, se accettiamo l'idea che la vita non è disponibile per il soggetto che la vive ma è disponibile per lo Stato, siamo all'inizio della riapertura di un'avventura storico-filosofica che consideravamo tramontata, quella basata sull'idea dello Stato etico, quello che dice al cittadino cosa deve pensare, cosa deve fare, a quale criteri e modelli di vita si deve uniformare, da che cosa deve farsi schiacciare. Siamo di fronte a tale prospettiva. Se la vita è indisponibile, noi teorizziamo che il libero intendimento del cittadino deve farsi schiacciare da un'autorità superiore e questa non può essere che quella dello Stato e della sua legge. Non lo accettiamo. Una norma di questo tipo non può essere accettata non può essere accettata sotto il profilo filosofico, storico e politico. È una norma pericolosissima! Io inviterei chi ha inventato questa formula della vita indisponibile a dichiararlo, perché mi piacerebbe vederlo in faccia. Chi l'ha inventata? Da dove viene fuori?

L'alleanza terapeutica, infatti, così come la maggioranza l'ha delineata, è totalmente asimmetrica: non è alla pari tra il paziente il medico, è un'alleanza tutta sbilanciata dalla parte della potestà del medico di prendere delle decisioni nel momento in cui il paziente non le potrà più prendere. Vi rendete conto che dentro questo nocciolo c'è l'impossibilità della vostra legge? Voi fate una legge sul testamento biologico che impedisce il testamento biologico, perché, se stabilite che il medico, alla fine, ha l'ultima parola, è come se ci diceste che esserci pronunciati non è servito a nulla. Ed è per questi motivi che siamo contrari alla formulazione dell'articolo 1.

il consenso informato ed un forte richiamo anche alla Costituzione. Il mio voto di astensione, e quello di altri colleghi, è coerente con l'impegno che c'è stato ed è anche di apprezzamento per il metodo di confronto che ne è seguito; spiace però che tale metodo di confronto sembra essersi esaurito con questo articolo 1 e con l'articolo 2, e che non sia proseguito in Commissione. l'auspicio che esso possa proseguire, magari nelle prossime ore in Aula, per rendere questa legge migliore e non per peggiorarla ulteriormente, come si è tentato di fare, come ha detto benissimo la collega Bassoli, con questi ultimi voti dell'Aula.

1. Votiamo a favore di una norma che fa una ricognizione dei principi su cui si basa, in un ordinamento

che si riteneva fossero assolutamente condivisi dalla nostra comunità nazionale, che discendono direttamente dalla Carta costituzionale e che sono sempre stati pacifici e non controversi. Poiché lo sono diventati

i valori di civiltà su cui si fonda la comunità che ha dato vita ad una Costituzione, di cui tutto si può dire tranne che enuncia valori negativi. La Costituzione, per principio, nel suo DNA enuncia valori positivi, traccia norme di principio, norme programmatiche e precettive, ma tutte in positivo e tutte rivolte a promuovere l'esistenza umana e mai a negarla.

di una persona incapace di intendere e di volere e che, in forza del combinato disposto di questo principio e di una non meglio definita interpretazione dei princìpi costituzionali,

anche il diritto alla riservatezza e al dolore si conchiudeva in maniera perfetta e senza bisogno di particolari

del patrimonio culturale e scientifico di questo Paese dall'entrata in vigore della Costituzione ai giorni nostri. Non dice nulla di più e nulla di meno, non incide sulla libertà dell'individuo, ma ne traccia i contorni secondo i valori

di sofferenza da parte di alcuni nostri amici del centrosinistra, su questa legge non abbiamo posto alcun obiettivo di ordine politico: riprenderò poi

quella che deve essere un'opera meritoria svolta da parte dello Stato, e in modo particolare del Ministero della salute, perché questi pazienti vanno assolutamente assistiti. Diremo poi che avete

personalistica, ma lo è anche in rapporto alle esigenze di una società. Non abbiamo fatto una Costituzione esasperata sull'individualismo: le culture

con le seguenti: «impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita»

di questa legge, quindi si tratta di un consenso anticipato. Inoltre, per rispondere brevemente al collega Pardi, sicuramente esiste un'alleanza terapeutica un'alleanza terapeutica che, ad una prima lettura, può apparire sbilanciata a favore del medico nei confronti del paziente. Io credo però che questo non sia assolutamente vero. Il concetto di alleanza terapeutica parte in maniera assolutamente paritetica nel rapporto fiduciario medico-paziente. È chiaro che, per determinate scelte, l'ago della bilancia si sposta verso il medico fondamentalmente perché, per poter applicare determinate dichiarazioni anticipate di trattamento che vengono fatte anni o decenni prima rispetto al momento in cui vengono messe in

che il cittadino - che a quel punto è diventato paziente - si trovi nelle condizioni di poter dare corso alla propria dichiarazione anticipata di trattamento, onde evitare di incorrere

con tutte le loro motivazioni, noi siamo convinti che debba rimanere un atto fuori della legalità perché nessuno deve poter decidere della vita o della morte di un altro individuo. Parallelamente - e questo è ancora più importante, per certi versi - bisogna garantire che su nessun individuo vengano compiuti gli atti di accanimento terapeutico che credo possano essere considerati addirittura peggiori rispetto all'eutanasia, perché obbligano ad una vita che non è più vita e costringono l'utente, il paziente, il cittadino - chiamiamolo come vogliamo - a subire degli atti assolutamente spropositati. Ritengo che sia fondamentale nell'impianto della legge che tutti questi concetti siano esplicitati già nell'articolo 1. Questo è il motivo per cui la pietra miliare è il voto a favore dell'articolo in

la Presidenza si è perfettamente resa conto che vi era stata un'incomprensione all'interno di tale Gruppo e ha ritenuto di dover adottare un metro di elasticità perché

sono preclusi gli emendamenti da 1.279 a 1.300, che tendono a modificare esclusivamente la rubrica dello stesso articolo,

Presidente, di emendamenti all'articolo 2 ne abbiamo presentati molti: alcuni cercano di proporre delle modifiche ragionevoli, altri di ridurre il danno

con il consenso informato si cerca un po' di coprire un danno che ormai é stato fatto.

Ai minori, agli interdetti, agli incapaci il consenso non è richiesto o, comunque, non interessa sapere come la pensavano e come la pensano, soprattutto quando c'è la situazione di pericolo di vita.

l'obiettivo di negare, svilire e annientare il significato del fare una legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Non è, insomma, l'uomo, la donna, la persona o l'individuo al centro di questa legge, sono l'autodeterminazione e il consenso informato che viene richiesto alla persona, ma altro. In altre parole, anche l'articolo sul consenso informato è

Interverremo, comunque, soprattutto come delegazione radicale, in corso d'opera e in corso di votazione degli emendamenti, anche se ci rendiamo ben conto che purtroppo il contingentamento voluto dai Gruppi e dal Senato

Spero che non sia così nel prosieguo della discussione. Temiamo, però, che questa piega e questa volontà di liberarsi al più presto possibile di questo dibattito sul testamento biologico

cui si prescrive che nessun cittadino può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria volontà se non per espressa previsione di legge e comunque nel pieno rispetto della propria dignità.

la questione del consenso informato non è stata regolata all'interno della dinamica tra medico e paziente. Addirittura il primo codice di deontologia, risalente al 1954, non prevedeva di fatto il consenso informato e solo in quello del 1989 la richiesta del consenso è diventato un vero e proprio dovere del medico, è apparsa per la prima volta la figura del fiduciario e si è

che un padre amorevole possa disporre della vita del figlio così come potrà disporre della propria:

*(PD)*. L'emendamento 2.22 riprende una formulazione di un gruppo di filosofi morali, tra cui i professori Semplici e Vigna, che tendono a costruire casi di eccezione e a far valere la volontà paziente e il diritto al rifiuto delle cure: ciò è

naturalmente del consenso informato: senza ripetermi nel ripercorrere e sottolineare l'importanza di tale conquista per i pazienti, vorrei evidenziare come il consenso informato copra l'interno vita del soggetto, garantendo il diritto di uscita dalle terapie e il rifiuto delle cure. Stiamo parlando di un concetto che vede il paziente protagonista delle proprie scelte e che risponde a una fondamentale e chiara volontà relativa a se e a quali cure sottoporsi. Naturalmente, abbiamo due o tre punti più sensibili e riteniamo che il consenso informato, a nostro parere, vada subordinato solo alla legge fondamentale dello Stato e, più precisamente, all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

si richiama la chiarezza sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla natura, sui benefici e i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, senza trascurare le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. Tutto naturalmente deve essere presente sulla cartella clinica. Tra i pazienti, colleghi senatori, vi sono anche - non dobbiamo dimenticarlo - i minori, i quali hanno diritto a dire la propria opinione, per cui bisogna prevedere il diritto da parte dei genitori e degli esercenti la potestà di accordare o rifiutare il consenso al trattamento medico dei minori, ascoltando però il minore e cioè considerando i suoi desideri e le sue richieste. **Saluto finestra"). Rivolgo un saluto agli studenti del Liceo classico di Casarano, in provincia di Lecce, presenti in tribuna in occasione della loro visita

su di sé e sul proprio corpo. Tali diritti sarebbero inevitabilmente violati dal carattere non vincolante, ma semplicemente orientativo di questo rifiuto. Pertanto, l'esclusione della vincolatività delle scelte individuali in ordine alle terapie e ai trattamenti da accettare e alla stessa inviolabilità del corpo priva del tutto il soggetto del diritto all'autodeterminazione e alla dignità personale, intesa quale divieto di uso e di strumentalizzazione della persona per fini che la trascendano.

informato nel caso di soggetto che si trovi in stato di incapacità legale assoluta o relativa. traduce, a mio parere in maniera più completa e meglio articolata, quanto già contenuto nel comma 6, prevedendo le varie possibilità

gli stessi obiettivi senza ricorrere alle procedure complesse che determinano l'interdizione e l'inabilitazione, anche in questo caso prevedendo la rappresentanza

**Il Senato non approva.**

che passa così inosservato e fa *pendant* con l'emendamento presentato all'articolo 1, pone una questione che aleggia in quest'Aula e che nessuno ha il coraggio di affrontare in modo chiaro. Io chiedo al relatore, al Presidente della Commissione e al Governo: se un cittadino capace di intendere e di volere di volere rifiuta il trattamento sanitario e il medico sa che quel rifiuto porta alla morte, il medico può imporre? Questa è la domanda a cui io chiedo umilmente risposta al relatore.

fondo. Se avessimo voluto giocare con il Regolamento del Senato, noi oggi avremmo potuto presentare un emendamento per inserire emendamento per inserire nella legge la seguente norma: se un cittadino capace di intendere e volere rifiuta la cura, i medici possono imporgliela.

allora ne fate solo una questione temporale, quando rifiutate che nel testamento biologico e nella dichiarazione anticipata

se lo scrive qualche tempo prima, glielo neghiamo? La sostanza del diritto è indisponibile, non cambia: mi dispiace che sia assente il professor Pera, perché quando affermate - com'è comprensibile - che, davanti ad un cittadino che consapevolmente chiede di non subire quel trattamento sanitario, non si può fare nulla, di fatto ammettete che quel diritto è disponibile. È notorio il caso di quella cittadina alla quale fu preannunziato che, se non avesse accettato l'amputazione della gamba,

Posso anche non essere d'accordo, ma tirate giù il velo: non potete continuare ad enunziare principi, quando sapete che abbiamo quest'impossibilità di fatto: non possiamo imporre il trattamento sanitario. Ecco perché il senatore Nania ha presentato l'emendamento 2.11: preoccupato di questo, sostiene che il paziente può soltanto esprimere parere contrario, perché si rende conto che, nel momento in cui il paziente

verità: in quel caso, il diritto alla salute era - ed è - più importante di quello di rifiutare la cura,

l'imposizione, perché tradireste la sostanza dell'articolo 32 della Costituzione. Ecco perché indirettamente, caro collega Nania, la ringrazio:

il senatore Procacci ha toccato un punto importante della nostra discussione, che tornerà in altri articoli, anche quando parleremo di vincolatività delle DAT. ha messo sullo stesso piano la situazione nella quale il paziente è del tutto cosciente, quindi può esprimere fino in fondo la propria libertà, con il caso nel quale, invece, queste situazioni si presentano in un momento altro rispetto a quando vengono fatte le dichiarazioni, e ha annullato o svalutato il senso e l'importanza della temporalità. Ci ha detto: è solamente un problema di temporalità. Guardi, senatore Procacci, che in quella temporalità che lei così sottovaluta passano problemi di ordine non solo filosofico, ma che fanno riferimento alla vita e all'esperienza di ognuno di noi, e dunque fondamentali. Credo che in Aula molti siamo genitori e sappiamo di aver compreso il senso di esserlo solo dopo che un determinato avvenimento è accaduto. Prima potevamo solo immaginarlo. Credo che in Aula, per una ragione anagrafica, molti di noi hanno avuto la sventura di perdere un genitore. Sappiamo che abbiamo compreso cosa questo significa solamente dopo che ciò è avvenuto. Noi non possiamo, come se nulla fosse, far passare una concezione programmatoria e deterministica dell'esistenza per cui in un dato momento precedente è possibile prevedere qualsiasi cosa. Guardi che per molti di noi la vita rimane un mistero fino all'ultimo giorno, e anche per chi non ha fede e non crede ed è intimamente liberale il futuro deve rimanere aperto. Ci deve essere almeno un piccolo spiraglio affinché tante teorie costruttivistiche che sono state applicate in maniera fasulla alla società non vengano applicate ora nell'ambito antropologico. È per questo che quella dichiarazione, quel concetto di alleanza terapeutica che fa tanto ridere alcuni in Aula e che è stato sbeffeggiato è invece al fondo della nostra proposta. Noi prevediamo che in questa legge ci sia quel dialogo e concepiamo le dichiarazioni anticipate come la possibilità di proseguire un dialogo anche nel momento in cui il paziente non è più presente con tutta quanta la sua intenzione. È questo il motivo per cui quella temporalità che lei così tanto svaluta è invece per noi così importante. Ed è su questo concetto che noi, all'interno del nostro Gruppo, siamo riusciti a riunire la gran parte dei cattolici e dei laici. Non è una ipocrisia. Non è una ipocrisia. È il modo per non passare ad un determinismo antropologico che, di fatto, leverebbe alla vita non soltanto ogni mistero ma anche ogni contraddizione. E la contraddizione è la libertà alla quale i laici non vogliono mai rinunziare. Ringrazio per le spiegazioni date, ma il mio emendamento è molto più semplice e dice cose molto più semplici. L'emendamento 2.11 innova il comma 1 dell'articolo 2 della proposta Calabrò. parte dal punto di vista che l'articolo 32 sostiene che la Repubblica tutela la salute. Quindi, la Repubblica - tanto per capirci il medico, l'apparato sanitario, il sistema

La Repubblica pensata dai Costituenti agevolava e favoriva ed ha una posizione principale nella tutela della salute. Il paziente, se non è d'accordo,

Ha ragione perché mi è stato segnalato dalla senatrice Mongiello che c'era qualcuno che stava votando per altri; per questo motivo ha ragione.

il seguente: «4-*bis.* Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario». È un principio chiarissimo: stiamo parlando di persone consapevoli e del diritto di ciascuno ad accettare o non accettare le terapie sanitarie, salvo i casi previsti dalla legge. Dire di no a questo emendamento significa, in realtà, svelare un'ipocrisia che è stata magnificamente definita dal collega Procacci.

con l'emendamento 2.64, che riguarda sempre la questione del consenso informato, proponiamo, e vorrei l'attenzione dei colleghi su questo, un esplicito riferimento all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che è già stato citato.

Ci sono dei soggetti che vengono completamente esclusi della possibilità che anche per loro valga il consenso informato. Con questo emendamento, in caso d'interdizione, nei casi in

la cui decisione avrà comunque lo scopo esclusivo di rispettare, in tutti i casi, la volontà espressa dall'incapace nelle forme stabilite dalla legge, perché l'incapace, prima di diventare tale, potrebbe aver lasciato le proprie dichiarazioni anticipate di volontà che dovrebbero essere comunque seguite.

Presidente, questa norma che riguarda i minori e dunque il consenso al trattamento medico del minore esclude un'attenzione alla alla partecipazione del minore. Quando parliamo di sedicenni o di diciassettenni di fronte ad una circostanza critica, ci rendiamo conto di quanto questa trascuratezza sia rilevante, però va notato che anche per adolescenti o per bambini una forma di coinvolgimento è necessaria. (testo 2) prevede che occorre ascoltare attentamente i desideri e le richieste del minore.

introduciamo un principio che rende ancora più vincolante l'espressione del consenso da parte del minorenne. Specifichiamo e aggiungiamo che quando il minore ha superato l'età di 16 anni,

di cui al presente comma, il consenso non è valido fino a decisione del giudice tutelare. Questo ragazzo di 16 anni deve avere la possibilità di far sentire il proprio consenso, che deve avere un peso e che non deve essere considerato una mera dichiarazione che resta agli atti.

nulla dice di nuovo rispetto a come oggi è normato il consenso informato nella pratica clinica e nell'attività degli ospedali? A me pare, ed è la ragione per la quale mi sento di dover richiamare l'attenzione dei colleghi, che sia soprattutto un modo per aprire una contraddizione nella legge. È forse uno specchietto per le allodole o il coronamento beffardo di una legge che, in realtà, è stata pensata e voluta proprio per ottenere la negazione del principio del consenso informato. È per questo, semplicemente, che voteremo contro

agli amici del centrodestra e, se avrò tempo, lo vorrei illustrare nel corso di altri interventi. In questi mesi, in Germania è stata presentata una legge di pochissimi articoli;

predicava fino a ieri l'eutanasia, avere altrettanta libertà in quella parte del Parlamento.

Mi rivolgo proprio ai senatori Cosentino ed Astore, con cui ci sono stati confronti importanti in Commissione. Certo, quello del consenso informato di per sé non è un principio innovativo: ciò è assodato, collega Cosentino.

a cui nessuno può sottrarsi, ed è vincolato a forme precise, pertanto non può essere interpretato. Esso non viene in aiuto dei medici; anzi, va a favore dell'approfondimento vero che il paziente deve avere e che non può essere affidato alla frettolosità o all'incompiutezza di un modulo che, proprio nell'emergenza dell'intervento sanitario,

Questa è una proposta che vuole tutelare maggiormente la volontà del paziente che versa in uno stato d'incapacità di accettare o rifiutare un consenso. Nella legge non si dice in modo chiaro, qualora il soggetto sia in uno stato d'incapacità, chi interviene in sua vece. Si consideri che siamo siamo sempre nell'ambito del rispetto del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione. Per questo, noi firmatari di questa proposta emendativa riteniamo che debba essere specificato come la struttura sanitaria e il medico debbano comportarsi.

importante che sia vincolante la volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In assenza di questa chiara volontà, bisogna attenersi a quanto manifestato al fiduciario nominato secondo la legge, o a quanto manifestato dal fiduciario nominato secondo l'articolo 6 di questa legge. Solo in mancanza di questi due elementi, il consenso e il dissenso al trattamento sanitario è espresso dall'amministratore di sostegno o dal tutore e, in mancanza, nell'ordine, dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dai figli, dal convivente

È previsto, infine, il ricorso al giudice tutelare se nessuna di questa ipotesi venga a realizzarsi. Signor Presidente, su questo emendamento, visto che votiamo soprattutto la vincolatività

Signor Presidente, devo ammettere che, se le correzioni previste su questo articolo verranno mantenute, tali modifiche troveranno non solo il mio pieno consenso, ma anche la mia piena soddisfazione. Tutti conoscono le mie forti perplessità sull'apertura nel nostro ordinamento all'istituto delle DAT, un istituto che poggia le sue basi sull'astrattezza del dichiarare oggi per allora. Non siamo stati noi, e non intendiamo esserlo in futuro, l'organo che si pone come interprete delle norme. Tale compito lo hanno già svolto impropriamente quelle parti della magistratura che, con varie sentenze, ci hanno condotto oggi fino a questo punto.

BIANCONI *(PdL)*. Tale legge andrà a modificare irrimediabilmente il nostro costume nei prossimi anni e determinerà una svolta nella professione medica e nelle pratiche dell'assistenza. Sarà solo il tempo a dirci se le norme che stiamo scrivendo non apriranno la strada ad una dilatazione del consenso informato nelle DAT. Infatti, se si interpreteranno queste ultime sulla scorta del consenso informato, le DAT finiranno per diventare obbligatorie. Ma, visto il clima del dibattito, ci siamo cimentati nella stesura di una DAT, che definiremo *light*, la quale garantisce i principi della Convenzione di Oviedo nel prevedere la possibilità, da parte del paziente, di esprimere desideri che il medico prenderà in considerazione; quindi desideri di cui terrà conto il medico quando opererà, sempre in spirito libero ed indipendente, mosso dall'unico intento di tutelare il bene del paziente. Questo perché quella del medico è una professione etica prima ancora che scientifica. Ho forti perplessità sulla previsione che la DAT assuma rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto sia in stato vegetativo e quindi non più in grado di intendere e di volere; dal coma allo stato vegetativo il soggetto non è mai in grado di intendere e di volere. C'è quindi il rischio che la norma possa essere interpretata da diversi soggetti (tra cui i magistrati) nella richiesta di accertare una tempistica per determinare il passaggio dalla reversibilità all'irreversibilità, oppure - ma spero che nessuno lo pensi - nella richiesta di estendere eventualmente questa norma anche a situazioni cliniche diverse dallo stato vegetativo, le quali vedrebbero la mia totale contrarietà. Potrei eventualmente ripensare al mio voto negativo se il testo fosse fortemente emendato sui punti precedentemente esposti e se si ci sarà una totale blindatura del concetto di idratazione ed alimentazione, così come previste nel testo Avevo aggiunto anche ventilazione, perché aria, acqua e cibo sono tutti funzionali al mero sostentamento vitale. Acqua e cibo, come sostentamento vitale, erano alla base del decreto condiviso dal ministro Sacconi e dall'intero Consiglio dei Ministri e da me - oggi, come allora - pienamente approvato. Per questo, sono contrarissima ad aperture che prevedano situazioni eccezionali o a porre come limite l'assorbimento. Su questo punto, la blindatura deve essere assoluta e determinata,

Presidente, anche se siamo restati in pochi, spero soprattutto che chi è andato via utilizzi la notte per riflettere e arrivare qua domani

e, soprattutto, si negherà l'evidenza e ciò che la scienza e la medicina sanno, dicono e scrivono, secondo quanto è documentato ovunque nel mondo. L'idratazione e l'alimentazione artificiali sono trattamenti medici: con quest'articolo 3, invece, neghiamo

delle persone con disabilità, sosteniamo appunto che l'idratazione e l'alimentazione artificiali, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale, fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita che non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Con quest'articolo, mettiamo la pietra tombale sul significato profondo che aveva il varo di una legge sul testamento biologico: certifichiamo che alcuni trattamenti sanitari sono obbligatori, contro il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, e andiamo contro la logica e contro quanto sta scritto in qualsiasi manuale universitario di medicina o in qualsiasi documento che parla della nutrizione e

non soltanto è da considerarsi a tutti gli effetti un trattamento medico, fornito a scopo terapeutico o preventivo, ma che - come tutti i trattamenti medici ha indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati e la sua attuazione prevede il consenso informato del malato o del suo delegato, secondo le norme del codice deontologico. Se diciamo, invece, che per quanto riguarda il soggetto incapace di esprimere quel consenso tutto questo non vale più, allora la domanda è: a che serve fare la legge sul testamento biologico? Qualche mese fa, qualche anno fa, il punto del contendere era la respirazione artificiale;

e a votare un testo che corrisponda a quello che succede nel resto del mondo e anche attualmente nei nostri ospedali, dove un medico non può nutrire

con questa legge, invece, noi lo imponiamo. Quindi, l'appello è che la notte porti consiglio e che domattina ci svegliamo un po' meno presi dalla ideologia e un po' più presi dalla razionalità.

Credo si debba tornare sul titolo di questo terzo articolo, perché forse vi è un errore di stampa: più che contenuti e limiti bisognava intitolarlo: «Limite dei contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento». Qui dentro vi è una lunga lista di tutto ciò che non ci può essere, a partire dall'elemento fondamentale per ciò che attiene ad un testamento, cioè la volontà dell'individuo che esprime, non i propri orientamenti, ma appunto i propri desideri arrivati alla fase finale della propria vita. Non mi soffermo su quanto già ha ricordato poco fa la senatrice Poretti. Ci tengo però a mettere un'altra volta agli atti che il costituendo partito del Popolo delle libertà ha recuperato pienamente non soltanto il concetto di Stato etico, ma anche quello di Stato sovietico. Infatti, voi prevedete

alla senatrice Poretti, a me, al senatore Paravia e alla senatrice Amati perché abbiamo pronunciato nei nostri interventi, negli ultimi mesi, i nostri testamenti biologici e quindi ci siamo salvati (colgo anzi l'occasione dei microfoni di Radio radicale per invitare gli italiani ad avvantaggiarsi, perché questa legge non sarà fortunatamente retroattiva),

circa l'attestazione della volontà dell'individuo. Tutti i nostri emendamenti vanno non nella direzione ottimistica della senatrice Poretti, perché abbiamo capito ormai che la ragione non alberga più qui, almeno per le prossime 48 ore, ma per cercare di limitare quanto più possibile i danni di questo testo di

né un regolamento sovietico né etico. Certamente, invece, è un convincimento che ci siamo creati anche da un dibattito approfondito svolto in Commissione, in un confronto costante con i colleghi. I miei emendamenti sono soppressivi per una parte, e per un'altra correttivi da un punto di vista formale per errori reali che si erano registrati: è sufficiente parlare di ASL e non di ASL regionale e quindi verrà eliminata la parola regionale. Ma vi è soprattutto un emendamento soppressivo sostanziale, tra l'altro presentato anche dai colleghi radicali, che sopprime il comma 3 dell'articolo 3; lo si fa per una maggiore chiarezza ed incisività, esattamente per il motivo per cui probabilmente era stato proposto e scritto in questa sede. Ma si determinava certamente una confusione importante poiché, come vediamo nell'inizio dell'enunciazione del comma, non era richiamato il suo riferimento alla dichiarazione anticipata di trattamento, ma poteva indubbiamente confondersi anche con quanto già precedentemente affermato nell'ambito del consenso informato. Ma per ciò che attiene ai contenuti ed ai limiti delle DAT

un accoglimento di quella che ci è sembrata una giusta riflessione, anche nella rimodulazione generale, approvando emendamenti che sono il frutto dell'intensità del dibattito, non solo nel confronto con l'opposizione ma anche nell'ambito della stessa maggioranza,

con serenità, anche nel rispetto delle norme deontologiche, della scienza e della coscienza.

quindi escluse dalle dichiarazioni anticipate di trattamento, questo emendamento contempla una fattispecie di sospensione. Se, infatti, il fiduciario è l'unico soggetto che è autorizzato a porre in essere le volontà espresse dal paziente e se queste non possono comunque mai configurare le fattispecie di omicidio, di istigazione al suicidio e di omicidio del consenziente, di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, *a fortiori* la sospensione dell'alimentazione può essere prevista solo qualora si verifichi l'irreversibilità della funzione propria di assorbimento e la perdita del metabolismo dell'individuo. Tale formulazione ammette sostanzialmente che il medico, in scienza e coscienza, possa porre in essere la sua capacità di giudizio. Infatti, per definire l'irreversibilità dell'assorbimento e la perdita del metabolismo occorre valutare ogni singola situazione e le peculiarità fisiche e cliniche della persona e del paziente. Tale valutazione deve essere soggetta ad una decisione, non solo del medico, ma anche di un collegio medico, in modo da cercare una sintesi scientifica

ma, finora, salvo qualche impegno preso nel corso di trasmissioni televisive da parte di qualche Ministro, che aveva promesso la convocazione di un tavolo tecnico-politico che coinvolgesse i sindacati, l'azienda e lo stesso

*(PD)*. Signor Presidente, come sicuramente i senatori presenti in Aula sapranno, nel mese di giugno a Pescara si terranno i Giochi del Mediterraneo. Da quando esiste questa competizione sportiva, lo Stato di Israele continua ad essere escluso per il veto imposto dai Paesi arabi.

porre la questione dei documenti relativi alla Conferenza di Durban 2, laddove si vuole equiparare il sionismo al razzismo. Inoltre, l'Italia è storicamente uno dei Paesi del Mediterraneo più vicini al mondo arabo, tanto da avere anche lanciato un piano Marshall in favore dei palestinesi. Quindi, l'Italia

grazie all'inclusione del territorio, ma non al riconoscimento della sovranità della comunità turca nel Nord - li ha esclusi dalla possibilità di essere rappresentati anche dal punto di vista politico e amministrativo all'interno dell'Unione europea, è stata fatta annusare loro la possibilità di diventare cittadini europei, attraverso il "Piano Annan" del 2004, salvo poi prendere la parte della popolazione greca.

Perduca, certamente lo sport per la sua tradizione e per le stesse origini di tutti i giochi, a cominciare dalle Olimpiadi, è sempre stato interpretato non solo come competizione sportiva leale, ma anche come occasione di pace e di incontro:

La seduta è tolta